nuova finestra"). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

La Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 27 ottobre. Nella seduta pomeridiana di oggi e nella seduta antimeridiana di domani proseguirà la discussione del disegno di legge sulle segnalazioni di reati o irregolarità nel lavoro pubblico o privato. Le dichiarazioni di voto sul provvedimento avranno luogo domani alle ore 11. Restano confermate, nella seduta pomeridiana di domani, le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri sul Consiglio europeo del 19 e 20 ottobre e il sindacato ispettivo nella seduta antimeridiana di giovedì 19 ottobre. I lavori della prossima settimana saranno interamente dedicati all'esame della riforma della legge elettorale con sedute uniche, senza orario di chiusura, a partire dalle ore 11 di martedì 24 sino a venerdì 27 ottobre, se necessario. La Presidenza potrà disporre sospensioni in relazione all'andamento dei lavori. La votazione delle eventuali questioni incidentali avrà luogo alle ore 17 di martedì 24 ottobre. Il termine per la presentazione degli emendamenti è stabilito per le ore 13 di lunedì 23. Il calendario potrà essere integrato con le comunicazioni del Presidente, ai sensi del articolo 126, commi 3 e 4 del Regolamento,

ho già fatto presente in Conferenza dei Capigruppo come la calendarizzazione forzata in Aula della legge elettorale, a meno di una settimana dal suo incardinamento in Commissione, rappresenta una violenza istituzionale di inaudita gravità. Di fatto, viene impedito al Senato di esaminare la legge elettorale e cioè la legge parlamentare più importante per la democrazia del nostro Paese. Questo avviene dopo un'altra forzatura molto grave, operata alla Camera con un intervento a gamba tesa del Governo che ha posto la questione di fiducia su una materia, che - ripeto - è per sua per sua natura squisitamente parlamentare. Ciò avviene anche a pochi mesi dalle elezioni, in un periodo in cui ancora più gravi risultano le prevaricazioni nella definizione delle regole del gioco da parte di alcuni giocatori, grossi e potenti, a danno di altri.

Presidente, lei conosce perfettamente l'articolo 72 della nostra Costituzione, il quale - lo voglio leggere qui testualmente «La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa».

e giustamente qualcuno l'ha definito un colpo di mano. Cosa accade ora? Anche in Senato ci troviamo di fronte a forzature che riteniamo gravi.

voluto che, questa volta, sul disegno di legge elettorale ci fosse una capacità di discernimento, di scelta, e non solo un badare ai propri interessi da parte delle coalizioni o delle finte coalizioni che si mettono in piedi pura convenienza. La lungimiranza e il voler bene al sistema democratico avrebbero dovuto in qualche modo indurre a un

Questa legge c'è e consente agli italiani con le pensioni al minimo, ai 17,5 milioni a rischio povertà, ai 9 milioni

a inizio 2017, ci ha indicato uno strumento che garantiva il diritto dei cittadini di scegliere i loro rappresentanti e anche la governabilità, perché sopra il 40 per cento di consensi consentiva una maggioranza adeguata per governare. Ma a quel punto la legge non è stata più accettata da lor signori perché, mondata dalle schifezze incostituzionali, non piaceva più, quasi fosse quello l'obiettivo. Chiaramente questa legge consentiva un Governo a 5 Stelle, con un programma per la prima volta votato dai cittadini. E questo non si poteva accettare: il Governo dell'unica forza politica che non accetta compromessi con i criminali.

è irrazionale; è una offesa all'intelligenza perché, da un lato, si predica il maggioritario e, dall'altro, lo si stempera con il proporzionale trainando il voto sulla persona con il voto di lista. In questo modo i cittadini non sanno più che

vuole oggi sapere, prima delle elezioni, che nessuno possa vincere. Allora, dal marasma emergeranno i veri soci del patto leonino, stipulato nel centro destra per votare Renzi, Berlusconi e Verdini e nel centro sinistra per votare Alfano, Renzi e Berlusconi. Vanno a caccia insieme per poi dare a questi due soggetti Signor Presidente, questa è una legge che non possiamo accettare nel merito ma, soprattutto, nel metodo e nell'*iter* che viene tracciato. Non è stata discussa alla Camera perché, con un sotterfugio, è stata rimandata in Commissione. Le audizioni e le discussioni svolte sul modello tedesco sono state date per buone su un modello che era totalmente l'opposto. Non sono state fatte le proiezioni che nessuno potrà governare, è perché i giornali ce lo hanno dimostrato con i conti alla mano, in quanto in Parlamento non si sono neanche preoccupati di fare questo tipo di simulazioni. Noi oggi queste cose le vogliamo fare, perché è un nostro diritto; perché senza questo diritto non siamo nel bicameralismo, e neanche nel

a un percorso predeterminato che, addirittura, forzava le prerogative della Commissione affari costituzionali. Tant'è che poi, in Ufficio di Presidenza della Commissione, ci siamo chiesti cosa potessimo fare, visto che eravamo Oramai era stata data la scadenza alla legge, neanche fosse una mozzarella acida. Che cosa potevamo fare? Non possiamo, poi, neanche organizzarci su questo perché ci hanno incastrato, tra il voto in

deciso. Il punto fondamentale è che le decisioni non vengono prese qui. Le decisioni sono già state prese. Lo abbiamo visto con quella manina che ha sbianchettato il testo alla Camera, il voto della Commissione e dell'Assemblea, modificandolo e restituendoci un testo che non è quello votato. M5S)*. Sorvolo appena su due questioni fondamentali. I figli del Porcellum hanno clonato il Porcellum nell'Italicum e quando quest'ultimo è stato mondato lo hanno disconosciuto e adesso ci stanno proponendo

autorizzi il Governo a violare la legge di contabilità, che prevede che la legge di bilancio sia presentata entro il 20 ottobre. Se prevediamo la calendarizzazione in Assemblea di quella che dovrebbe essere la sessione di bilancio ottobre, noi stiamo legittimando il Governo a fare scempio della legge di contabilità. Stiamo delegittimando la Commissione affari costituzionali nonché la Commissione bilancio,

Stiamo svuotando di senso queste Aule, stiamo dicendo che ormai l'Italia è stata sottratta, portata via ai cittadini che attendono invece il futuro da un Parlamento finalmente legittimo e da un Governo che affronta veramente i problemi. Lo vediamo da come, invece, è stato insabbiato il provvedimento per l'abolizione dei vitalizi. Il partito unico dei vitalizi, il partito unico del finanziamento ai partiti e delle sanatorie ai loro bilanci

la senatrice De Petris parlava di consapevolezza del voto da parte dell'elettore, del cittadino; io, per la verità, parlo di consapevolezza del voto di noi parlamentari. La legge elettorale, colleghi, è uno strumento di democrazia, ma è anche un provvedimento oltremodo complesso, che va studiato e approfondito perché si possa esprimere un voto con convincimento. Dovendo esprimere Dovendo esprimere un voto che regolamenta i principi di governo del mio Paese, io sento l'esigenza forte di dover approfondire la legge, di doverla studiare e di dover poi assumere una determinazione

anche se proviene da una forza politica diversa da quella alla quale io aderisco, ma devo essere convinto che ciò che sto votando

costituzionale a bocciare il provvedimento per incostituzionalità; facciamo un buon lavoro insieme. La legge elettorale deve essere fatta insieme, anche con il Movimento 5 Stelle. Facciamola bene, facciamola insieme. Poi, taluni possono anche non essere d'accordo, ma almeno facciamo salvo il profilo tecnico, la correttezza scientifica

ai cittadini. Ebbene, questo Parlamento non vuole abolire un privilegio, perché di questo si tratta, è inutile che lo nascondiamo: un trattamento di favore che consente, dopo quattro anni e sei mesi, di avere una pensione che un cittadino non vedrà neanche forse forse prima di morire. Dicevo, per non eliminare questo privilegio, è da settimane che facciamo audizioni. Per questo motivo, Presidente, chiedo che sia calendarizzata, già da giovedì mattina, la

che ha un'ampia condivisione in Parlamento (quando parlo di ampia condivisione mi riferisco a forze che fanno parte della maggioranza di Governo e a forze largamente rappresentative dell'opposizione), non si possa parlare di scorciatoie. Legittimi dubbi di costituzionalità ci possono essere, ma questa proposta risponde ai requisiti che la Consulta aveva fissato: liste brevi e collegi uninominali che consentono

Per quanto riguarda la questione dei vitalizi, menzionata poco fa, vorrei dire al senatore Crimi che le audizioni in 1a Commissione non sono state affatto inutili. Se i commissari del Movimento 5 Stelle le avessero ascoltate,

Presidente, è molto imbarazzante la discussione che si sta svolgendo in un'Assemblea che ha già discusso una legge elettorale dichiarata incostituzionale. Evidentemente non impariamo le lezioni e siamo abituati a vedere Presidenti del Consiglio, Ministri, Capigruppo che dicono una cosa e poi ne fanno un'altra.

della Camera, ha commesso, e in particolare a valutare la legge sugli orfani nel femminicidio, votando l'emendamento che evita che si possa assegnare effetto riparatorio...

sentire, sullo *ius soli*, questa orchestra dei vari Ministri, in cui uno dice che bisogna votarlo e l'altro che invece non è il momento. Noi vorremmo che quest'Aula si occupasse finalmente di questi due provvedimenti, quello che riguarda gli orfani del femminicidio e quello che riguarda lo *ius soli*, per assumersi delle responsabilità, anziché rincorrere in velocità una legge che avrebbe bisogno di maggiore ponderazione. A riprova di questo, signor Presidente, faccio presente solo una cosa, che non ha a che fare con i difetti di costituzionalità, ma con la fretta con cui si scrive. Viene riscritto, con una tecnica emendativa molto discutibile, il primo

c'era scritto («attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali»), questo vuoto è stato colmato con un'espressione che non ha molto senso, perché non si capisce come dovrebbe essere se non un unico turno elettorale, visto che non c'è più il ballottaggio e visto che siamo una nazione unica e una Repubblica che ha un unico turno elettorale. questo, per dire che queste leggi sono raffazzonate e che sui vizi di costituzionalità si guarda con troppa superficialità, perché poi saranno evidenti quando si pronuncerà la Corte e ci sarà un altro Parlamento: si ha uno sguardo corto. Io vorrei avere uno sguardo corto nel senso di fare in questa legislatura quello che possiamo fare

maniera indecente: beh, ci sono delle contraddizioni, ma che vuole? Era un compromesso: un pezzo l'ha voluto uno e un pezzo l'ha voluto l'altro. Questa è la legge elettorale. Doppio sistema, maggioritario e proporzionale? Un pezzo l'ha voluto uno e un pezzo l'ha voluto l'altro. I nominati e non le preferenze? Un pezzo l'ha voluto uno e un pezzo l'ha voluto l'altro. Con quale serenità si può discutere in quest'Aula? Io non ho votato l'Italicum, non ho questa macchia; ma chi ha votato l'Italicum dovrebbe riflettere sul fatto che vorrebbe e che pretende di farci votare per la seconda volta una legge incostituzionale.

Presidente, devo dire che prendo la parola con difficoltà, perché ho perso il filo di questo dibattito. Mi è sembrato che, a un certo punto, il dibattito prendesse la via dell'ostruzionismo, con vari parlamentari dello stesso Gruppo che prendevano la parola per proporre ordini del giorno diversi da

Vorrei ricordare al Senato che siamo a pochi giorni dall'inizio della sessione di bilancio. Vorrei ricordare al Senato che il Senato stesso ha deciso che giovedì di questa settimana noi non lavoreremo, perché dobbiamo lasciare il tempo - io credo legittimamente - ai parlamentari che intendono partecipare alle campagne elettorali in Lombardia e in Veneto.

In questa situazione, noi dobbiamo tener conto del fatto che l'Italia ha bisogno di una legge elettorale; ha bisogno, cioè, che venga evitato che tra pochi mesi gli italiani vadano a votare con due leggi elettorali molto diverse; il risultato di quel voto sarebbe certamente due Camere nelle quali sarebbero presenti due maggioranze diverse. maggioranze diverse. Abbiamo approvato un calendario che fa lavorare la Commissione affari costituzionali per una settimana; la Commissione si è già riunita oggi, ha approvato il suo calendario, ha stabilito il termine per le audizioni, per la discussione generale, per la presentazione degli emendamenti e il momento in cui si andrà a votare. Non sappiamo se il Governo deciderà di apporre la questione di fiducia o no; il Governo lo deciderà, ma questo dipenderà anche da noi,

Presidente, io penso che a ciascun senatore dovrebbe essere data la possibilità di parlare senza essere interrotto. *(Applausi dal

Parlano, invece, dei vitalizi, ben sapendo che la Commissione ha addirittura già determinato

Io voglio dire, signor Presidente, che sulla legge elettorale vogliamo una discussione che consenta di approvarla in un momento nel quale al Parlamento sono dati tempi determinati. Tempi determinati da decisioni nostre, perché il giorno in cui non verremo in Aula lo abbiamo deciso noi, e dalla concomitanza con la legge di bilancio. Questo vogliamo e questo chiediamo che l'Assemblea approvi.

inserire il testamento biologico tra le cose che dobbiamo fare in questo scorcio di legislatura. Sarebbe davvero molto bello se il Parlamento chiudesse questa legislatura

proprio perché siamo a fine legislatura, dobbiamo fare la legge elettorale. Peccato, presidente Zanda, che quell'Europa che lei tante volte richiama - gliel'ho sentito dire molte volte in questi quattro anni e mezzo di legislatura

in Parlamento vincerete, ma era già successo qualche tempo fa. Eppure, la storia dovrebbe insegnare qualcosa: anche quando avete fatto la riforma costituzionale, in Parlamento avete vinto. Avevate i numeri in Parlamento e anche in quel caso, come oggi, a colpi di maggioranza, avete cambiato la Costituzione. Poi però è successo un piccolo contrattempo che non avevate considerato: parlato il popolo sovrano, oltre al Parlamento. E il popolo sovrano ha clamorosamente smentito la vostra maggioranza che avevate costruito sulle riforme. Vedrete che finirà esattamente nello stesso modo: anche questa volta state imponendo, in questo caso un cambiamento di legge elettorale e non una modifica della Costituzione, a maggioranza e lo state facendo ricorrendo alla fiducia, peraltro mettendo il nome del Governo Gentiloni Silveri nel triste elenco di quei Governi che, per l'appunto, ricorsero alla fiducia per cambiare le regole del gioco, e lo state facendo a pochi mesi dalla fine della legislatura.

che anche la legge elettorale che state facendo molto probabilmente cadrà sotto la mannaia della Corte costituzionale e avrete contribuito sempre più a far sì che in questo Paese la considerazione dell'opinione pubblica verso le istituzioni repubblicane fosse peggiore di quella già drammatica che si è determinata in questi anni. Ma come fate a caricarvi questa responsabilità?

Come fate a non capire che siete voi i principali responsabili di quello che sta accadendo in tutti questi anni? Eppure avreste dovuto capire almeno la lezione

che un manipolo di eletti possa modificare le regole democratiche in questo modo. E voi davvero volete insistere su questo terreno? Davvero volete costruire questo tipo di meccanismo? Davvero, ancora una volta, presentate le liste bloccate? Davvero, ancora una volta, costruite un'ipotesi per cui la democrazia debba essere mortificata in questo modo? Fossi in voi, sarei molto accorto rispetto a quello che state facendo e sarei molto più attento molto più attento a quello che ha detto la cittadinanza di questo Paese nel corso di questi mesi e di questi anni. Il popolo sovrano ha parlato in maniera molto chiara e molto netta. Ha dato un messaggio molto chiaro e molto netto il 4 dicembre di qualche tempo fa: il fatto che lo abbiate dimenticato così velocemente e con l'arroganza di una maggioranza che è tutta qui, è tutta all'interno di quest'Aula parlamentare, ma non ha nessuna riscontro nel Paese reale, penso che lo pagherete molto, molto caro.

Anziché imporre la fiducia e sbianchettare qualche errore grossolano provocato dall'incompetenza di chi scrive le leggi, avremmo preferito poter discutere tranquillamente senza trovare scuse. Ricordo ancora quella notte trascorsa qui, il 22 dicembre 2015, con la Finocchiaro, poverina, piegata in due a dover incardinare l'Italicum per far contento Renzi, e si era nel

- vorrei rivendicare la possibilità da parte del Movimento 5 Stelle di approfondire la legge elettorale con le audizioni e attuare una una discussione animata, compiuta e puntuale in Commissione, come da quattro anni e mezzo stanno a gingillarsi sui vitalizi, perché il Partito Democratico non dice che non ha capito la sua stessa legge, che ha votato alla Camera ma qui invece ha bisogno di capire, che non capisce; sono dei "cretini", che non hanno compreso che devono lasciare il malloppo della pensione prima di garantirsi la poltrona per tornare qui dentro! *(Applausi dal

di fare un altro papocchio e far ridere il mondo con la terza legge elettorale incostituzionale.

votazione (\*)** Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato

Ci sono i responsabili anticorruzione dei vari settori e dovrebbero bastare quelli, i quali devono vagliare un minimo le segnalazioni, perché altrimenti non servono a nulla. Ipotizzare che qualunque cosa debba essere segnalata all'ANAC sarebbe come

di impedire all'ANAC di funzionare, se non su segnalazione, per cui l'ANAC riceverà un miliardo di segnalazioni del tutto inutili, e poi, se vorrà fare qualche azione specifica in modo arbitrario e discrezionale, potrà farlo. Credo che nessuno condivida questo

ci sia una sentenza di primo grado sfavorevole al segnalante. Vorrei sottolineare il fatto che indubbiamente il processo che può riguardare il segnalante si affianca all'altro procedimento, che è quello di verifica della fondatezza delle segnalazioni.

che non debba) averne conoscenza, ovvero fino alla chiusura delle indagini preliminari. Tuttavia, signor Presidente, lei sa meglio di me che l'articolo 111 della Costituzione (quello sul giusto processo) consente all'imputato di assumere mezzi di prova a sua difesa. all'articolo 111 che, unitamente all'articolo 25 della Costituzione, è il fondamento costituzionale delle indagini difensive. Per rappresentare la delicatezza della questione, che sempre l'articolo 111 della Costituzione, sia pure con riferimento alla fase del dibattimento, afferma che l'imputato non può essere condannato sulla base delle dichiarazioni di un soggetto che rifiuta di essere interrogato dall'imputato. Questo appartiene alla fase successiva,

in che modo un soggetto può assumere mezzi di prova a sua difesa, così come espressamente garantito dalla Costituzione all'articolo 111, se non conosce il nome della persona che ha svolto dichiarazioni accusatorie nei suoi confronti? Ella sa, signor Presidente - come credo sappiano tutti i signori senatori che la giurisprudenza della Corte costituzionale sul punto, con riferimento all'articolo 111, è sufficientemente chiara e afferma che, tra i mezzi di prova che possono essere assunti dall'indagato/imputato a sua difesa, sussistono anche quelli posti strumentalmente a dimostrare la falsità delle dichiarazioni - per le quali oggettivamente non vi sarebbe necessità di conoscere l'identità del dichiarante ma anche l'attendibilità del dichiarante. Mi chiedo, allora, signor Presidente, come si possa ritenere costituzionalmente legittimo questo inciso, che va a limitare pesantemente l'articolo 24 della Costituzione, il diritto di difesa, in specie e a fronte di quanto prescritto dall'articolo 111. Il senatore del Movimento 5 Stelle Crimi e gli che pure hanno verso il provvedimento una visione molto diversa, se si vuole, osando una categoria corrente, molto più giustizialista che garantista, si erano posti il tant'è vero che inserivano prima di tutto la possibilità del consenso (io accuso, ma acconsento a che venga svelata la mia identità), la qual cosa, secondo il chiaro disposto del comma 3 dell'articolo 1, non è assolutamente possibile. senatori aggiungevano poi che nel procedimento penale le dichiarazioni rese da un soggetto che non presta il consenso, e che quindi rimane anonimo, sia pure fino alla chiusura delle indagini preliminari, non erano di per sé sufficienti per il prosieguo procedimentale, in assenza di ulteriori autonomi elementi. Questo è corretto. È chiaro che potete votare questa norma, tanto una più una meno cambia poco, vi sarà la polemica sul punto, similarmente a quanto accaduto per il codice antimafia, vi cospargerete il capo di cenere e direte che proverete ad aggiustare la vicenda con un successivo intervento. La realtà di fondo, signor Presidente, è che questa piccola disposizione, che poteva essere tranquillamente pretermessa o quantomeno ammorbidita, seguendo la posizione proposta dal Movimento 5 Stelle, è in chiara violazione del diritto di difesa e del diritto al giusto processo, che - è inutile ricordarlo in sono diritti fondamentali della nostra Costituzione, considerati nell'ordinamento internazionale come diritti inviolabili. Il tutto equivale a dire: andate avanti in questa foga giustizialista;

l'obiettivo da raggiungere giustifica il mezzo con cui lo si raggiunge. Tutto questo fa strame del codice di procedura penale, e cioè di quel codice posto a tutela delle garanzie del più debole, che è, per l'appunto, l'imputato. Andate avanti,

davanti alla Corte costituzionale perché è asimmetrica non solo nei confronti della nostra Costituzione ma anche nei confronti del nostro ordinamento internazionale.

In un Paese democratico, la limitazione del diritto alla difesa è una delle questioni più gravi che si possano introdurre all'interno dell'ordinamento. Noi lo stiamo facendo con questo con questo articolo: stiamo creando le condizioni affinché i cittadini non possano difendersi rispetto ad accuse che possono essere infamanti e non giustificate da alcun fatto concreto. L'ho già detto nella discussione generale: questo è un provvedimento che potrà mettere in campo regolamenti di conti, attacchi a concorrenti, messe in discussione di posizioni all'interno della pubblica amministrazione semplicemente perché si dà fastidio a qualcuno e l'accusatore si crea una protezione successiva perché fa il delatore (la sostanza è questa). Di fronte a questa degenerazione della giusta lotta alla corruzione e ai comportamenti illegali nella pubblica amministrazione, noi diciamo di no, perché c'è sicuramente qualche altro metodo che consente di avere una pubblica amministrazione responsabile e rispettosa dello Stato di diritto, e dei cittadini convinti che per fare il proprio dovere

dell'articolo 1 esprime qualcosa che è avvicinabile al concetto della delazione, fenomeno antico

vale a dire Domiziano, gli riconosceva di aver contrastato e perseguito i delatori e la delazione.

alla rivelazione della sua identità anche la sorte del procedimento disciplinare attivato sulla base della segnalazione. Si tratta di una norma che produce un risultato oltre che paradossale anche ingiusto. Chi venisse incolpato sulla base di una segnalazione in un contesto in cui l'identità del segnalante sia indispensabile per la sua difesa, si vedrebbe probabilmente prosciolto sì, ma comunque sottoposto a un procedimento del quale gli rimarrebbe sempre e comunque ignota la scaturigine. Dice bene il senatore Buemi: non è possibile immaginare che non si dia la possibilità di difesa ad un soggetto che viene incolpato, ancorché nell'ambito di un procedimento disciplinare. Svetonio e non sono Domiziano. Però, come Svetonio e come Domiziano, mi oppongo

dal Gruppo perché non mi sento di votare né contro, né a favore; e ne spiego la ragione, che lei coglierà certamente meglio di me. Questa norma è in parte ridicola e in parte inapplicabile. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. La mia domanda è rivolta non a lei, signor Presidente, ma al relatore: come faccio a sapere che è necessaria, nel procedimento disciplinare per la mia difesa, la conoscenza dell'identità del segnalante? Non so nulla. L'identità del segnalante è coperta, c'è una notizia che mi riguarda e che ha dato luogo a un'iniziativa disciplinare e io devo chiedere l'identità del segnalante perché è necessaria alla mia difesa? Ci rendiamo conto che è una cosa assurda e impossibile? Come faccio io incolpato a pensare che l'identità del segnalante possa essere utile alla mia difesa? A meno che non abbia rivelato una notizia che riguarda tutti e due, per cui l'incolpato avrà

che non ha senso e che nessuno di noi riesce a comprendere? Figuriamoci quando dovrà essere applicata! di un legislatore è la chiarezza non solo della norma, ma anche della finalità che questa persegue. Siccome qui la finalità non si comprende,

voteranno contro questo articolo. Però, nel momento in cui lo dichiariamo, speriamo, sulla base delle considerazioni

qui sono state mosse considerazioni molto pertinenti in materia di rispetto della Costituzione. senatore Falanga il delatore è figura odiosa; ma, per quanto odioso sia il delatore nella Roma di Svetonio, mi si consenta di dire che altrettanto odiose sono l'indifferenza, l'insofferenza e (se posso usare questa espressione) la strafottenza di un'Assemblea parlamentare di fronte al diritto al giusto processo e al diritto alla difesa che finirebbe per

le abbiamo fatto notare che questo provvedimento non è mai passato per la Commissione giustizia. Lei ci ha detto che non era proprio così. Per noi che non facciamo parte di quella Commissione era esattamente così e la documentazione del fascicolo lo testimoniava. Credo che questa discussione imponga alla buona fede

i senatori della Federazione della Libertà voteranno, come hanno detto tutti i colleghi che mi hanno preceduto, in maniera contraria.

vi sono alcuni emendamenti che cercano nel loro insieme di circoscrivere l'applicazione di norme, la cui irrazionalità, con rischio di inapplicabilità e incostituzionalità, è stata ampiamente approfondita

previste tutele e sanzioni nei confronti di chi segnala irregolarità anche nel settore privato. Devo dire che in questo caso la norma è sempre più acrobatica e sempre più difficile da circoscrivere. I miei emendamenti tendono a circoscriverne l'applicazione. L'emendamento 2.202 chiede che le condotte illecite vengano segnalate entro sette giorni dal momento in cui il segnalante ne sia venuto a conoscenza, per evitare

chiede che queste segnalazioni siano fondate su elementi di fatto precisi e che comportino gravi violazioni del modello di organizzazione e

il che in via del tutto teorica va molto bene, ma in pratica significa incitamento alla segnalazione generica, verosimilmente inconcludente,

Trovo che l'articolo 2, intitolato «Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato», sia stato molto negletto all'interno di questa legge.

ci ha chiesto di recepire a proposito dell'antiriciclaggio, un articolo corposo dava una serie di indicazioni e di principi ai quali avremmo dovuto far seguire delle indicazioni operative, proprio nella direzione della tutela del segnalante; e stiamo parlando di privato. Ora, invece di fare passi avanti, con queste definizioni stiamo facendo passi indietro rispetto anche all'esistente introducendo un obbligo relativo «elementi di fatto precisi e concordati», che chiediamo al privato e non al pubblico, quand'è proprio in un certo tipo di privato che le segnalazioni si sono rivelate più importanti e rilevanti anche ai fini di un interesse collettivo. Ricordiamo che le banche

e qui viene introdotto nel privato, oltretutto in modo del tutto incoerente rispetto ai principi del modello organizzativo perché quest'ultimo riguarda l'organizzazione della prevenzione della corruzione. Chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate ha un suo percorso che riguarda la querela e i relativi procedimenti conseguenti alla stessa. Per questo l'articolo 2 è particolarmente

dare una struttura che sia certa e chiara e che fornisca indicazioni sia al privato, quindi all'azienda, sia al segnalante perché

come un fatto ancora esistente) abbiamo visto che negli Stati Uniti c'è addirittura un premio per i segnalanti, cioè per coloro che fondatamente segnalano. In realtà, nel corso della discussione alla Camera, il concetto del premio era stato superato

non è affatto superata la necessità di un fondo, tanto è vero che sono stati presentati ordini del giorno che chiedono al Governo di istituirne uno. Ora, io non capisco per quale ragione debbano essere accettati degli ordini del giorno quando qui

che si chiude con la certezza di recuperare risorse per dare quelle tutele che sono il contenuto e il significato principale di questa legge. Un altro aspetto che mi sta molto a cuore riguarda le clausole contrattuali di fedeltà e riservatezza. A fronte del prevalente interesse pubblico, sono nulle. Questo è il contenuto dell'emendamento 2.209 che io non ritengo superato dall'emendamento del relatore 2.0.200

anche rispetto all'articolo 1, si ritaglia una condizione particolare di non coinvolgimento in questa responsabilità di prevenzione della

la prevenzione della corruzione ci spinge a richiamare tutti i cittadini e a dare loro una tutela in modo del tutto contrario

in un'attività di delazione, ma nell'esercizio del loro senso civico con responsabilità; per questo ritengo non sia giusto ritagliare intorno a queste figure una sorta di area di liceità, di vincolo e di non coinvolgimento in questa responsabilità.

della presente legge, ove compatibili», cercando così di risarcire il grave squilibrio che, a mio avviso, c'è, tra la tutela nel pubblico e la tutela nel privato. Ricordo

Ricordo che cinque anni fa abbiamo introdotto una norma che mi piacerebbe fosse monitorata. In tutti i Comuni italiani è stato realizzato obbligatoriamente il piano anticorruzione. In ognuno degli 8.000 Comuni italiani c'è quindi un funzionario

denuncia la condotta illecita, siamo sul piano del reato, di un atteggiamento del privato e di qualcuno che approfitta all'interno dell'azienda. Non ci fermiamo però che la denuncia può essere fatta sulla condotta illecita o violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente.

rivolgo anche alla sinistra, che in un Paese civile e democratico, questa fosse la posizione del sindacato. Cosa fa il sindacato dentro un'azienda se non operare

Che titolo ha il singolo dipendente per mettersi a discutere della gestione o dell'organizzazione dell'ente, magari anche in forma anonima? se sia possibile introdurre la stessa clausola che è stata introdotta nell'accordo sulle banche, ossia che ciò avvenga secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, affinché in questo meccanismo il sindacato non venga totalmente totalmente scavalcato e anche delegittimato rispetto alla sua funzione. E non mi sembra una provocazione da poco. Poi naturalmente mi rimane da capire, ma vorrei sentirlo dal relatore e dal Governo, perché si passa dalla denuncia delle condotte illecite alla segnalazione di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, che mi sembrano due cose completamente diverse, ma che sicuramente comportano, all'interno dell'azienda, il pericolo di una gestione personalizzata, coperta dall'anonimato. Vi è il rischio

una questione generale: il nostro ordinamento ha già introdotto una disciplina generale sulla protezione del dipendente che segnala illeciti. Non è una novità:

Ovviamente si guarda alla modifica della responsabilità amministrativa degli enti privati che deriva da reati. Che cosa dice la norma, perché altrimenti rischiamo di capirci male? La disciplina prevede la responsabilità di enti, associazioni o privati, nonché di enti pubblici economici, per i reati commessi da alcuni soggetti nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Oggi interveniamo semplicemente con una definizione ulteriore, a tutela del segnalante, di quei requisiti e non sul quadro generale che è già

come funziona il sistema, ma non indica con chiarezza che cosa deve fare chi si trova in questa difficile e scomoda situazione, cioè una persona che nel suo lavoro è venuta a conoscenza di quella che gli sembra un'attività illegale,

2 istituisce nuovi obblighi per tutte le società e addirittura associazioni, anche prive di personalità giuridica, intervenendo sul decreto legislativo 8 giugno 2001,

che abbia segnalato qualche irregolarità nella pubblica amministrazione, anche se non c'entra nulla con l'azienda in cui lavora, ha diritto a tutele particolari per evitare misure che peggiorino le sue condizioni lavorative, anche di carattere organizzativo. Questo è quanto stabilito dall'articolo 1

che prenda un provvedimento che rende più gravosa la situazione lavorativa di un suo dipendente viene punito con una multa da 5.000 euro in sù

ma se non è in grado di dimostrare di aver preso le misure preventive necessarie (che sarebbero un piano annuale contro la contro la corruzione e la rotazione degli incarichi). Colleghi, notate bene che queste previsioni valgono anche per i tanti Comuni che hanno un solo dipendente. Questo unico dipendente, deve perdere tempo prezioso - durante il quale dovrebbe rendere servizi alla popolazione del suo Comune - per fare una relazione in cui spiega come previene attività di corruzione di cui egli stesso può essere l'unico autore, essendo l'unico dipendente.

ha commesso qualche illecito a vantaggio della società stessa, la società ne subisce le conseguenze ed è ritenuta essa stessa responsabile. Dunque, se colui che ha commesso questo atto non è il presidente sarà

istituendo, tra l'altro, uno o più canali che consentano ai soggetti indicati di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate. Tali canali,

attraverso il quale dimostrare di avere segnalato a questo dipendente che esiste il modo di denunciare irregolarità e, quindi, il modo di essere protetti. Una serie di adempimenti burocratici che produrranno montagne di carta ma per i quali non serve la copertura, perché tanto paga il privato.

se salta fuori che questi ha commesso una irregolarità e che si è dato da fare al di là del lecito, la società stessa ne è responsabile. Dunque, tutte queste associazioni dovranno dotarsi di queste strutture burocratiche, che alle grandi aziende, siccome hanno già

a realizzare un profitto, se è un'azienda di tipo commerciale o industriale, o a svolgere l'attività oggetto dell'associazione,

non potrà dare luogo ad alcun provvedimento contro chi l'ha fatta perché, se si segnala un fatto preciso, solo in quel caso si può ravvisare la calunnia e, alla lunga, questa persona sarà punita. La segnalazione generica, però, consentita dall'articolo 1, sarà premiata. Qui, inoltre, abbiamo anche la burocratizzazione burocratizzazione delle aziende private. E poi ci si stupisce se le aziende preferiscono il nero e preferiscono spostarsi in altri Paesi. Io propongo, dunque, non la cancellazione di questi obblighi,

che costano a chi le fa e il cui costo si riversa su chiunque goda dei servizi di questi enti, sia dal punto di vista monetario sia dal punto di vista di minori servizi prestati.

propongo che le condotte illecite vengano segnalate entro sette giorni dal momento in cui il segnalante ne sia venuto a conoscenza, per fare in modo

perlomeno si abbia una relazione immediata tra il momento in cui il segnalante viene a conoscenza dell'illecito o del presunto illecito o di qualcosa di molto generico descritto all'articolo 1

o anche un'altra - stava facendo qualcosa di irregolare contro la pubblica amministrazione; così si guadagna questa assicurazione contro qualsivoglia qualsivoglia provvedimento che lo possa danneggiare. Qualcuno dice che non può essere così, perché dovrebbe prima aver fatto la segnalazione e poi subirne le conseguenze.

un buon proposito, quello di tutelare quanti segnalano irregolarità della pubblica amministrazione ma poi il testo porta a una deriva che lo conduce da tutt'altra parte; facciamo in modo qua e là di di andare nella direzione suggerita dal titolo. Per ora faccio notare che, tranne quell'emendamento che per la verità ha cambiato pochissimo (ma sempre meglio di niente) l'articolo 1,

cosa che avrebbe dovuto essere fatta prima - sanzioni anche nei confronti di coloro che abbiano riportato responsabilità di natura penale per i reati di calunnia o diffamazione nell'ambito delle segnalazioni qui previste. Colleghi, questo è uno dei tanti problemi che emergono con questo disegno

prendere provvedimenti disciplinari nei confronti di un dipendente: dobbiamo prenderne atto; qualcuno potrà esserne contento, qualcun altro no, ma dobbiamo prenderne atto. Negli Stati Uniti per un dipendente che faccia una segnalazione

come funziona il diritto del lavoro e le sentenze, che a volte sono fatte, mio parere, in modo più consono a quello che dovrebbe essere il buonsenso, nell'interesse di tutti i lavoratori,

dell'interruzione del rapporto di lavoro. Sarebbe un modo per equilibrare; allora sì che vagamente si giustificherebbe l'introduzione di criteri che non sono del nostro sistema e della nostra legislazione. Introdurli in questo modo è veramente un obbrobrio che non tiene conto della realtà.

e non eccessivamente burocratica. Il problema di molte norme approvate in questa prestigiosa Aula, spesso con le migliori intenzioni, è che ci sono degli effetti secondari non voluti. Si vorrebbe imporre una serie di adempimenti che hanno l'idea di essere preventivi rispetto alla commissione di reati, ma qui, in realtà, non si tratta di provvedimenti preventivi alla commissione di reati, bensì di provvedimenti che si propongono di prevenire possibili ritorsioni a danno di chi forse segnala in modo del tutto generico delle irregolarità nella pubblica amministrazione. Tutta questa grande preveggenza, che peraltro se si usasse anche in altri settori forse farebbe prendere delle decisioni più responsabili, dimentica un fatto: che tutte le volte che si stabiliscono delle sanzioni di questo tipo, si impongono a tutti a tutti i soggetti, in particolare a coloro che non hanno alcuna intenzione né di commettere reati contro la pubblica amministrazione né di attuare misure ritorsive contro chi segnala eventuali reati nell'ambito della pubblica amministrazioni,

Ma ci rendiamo conto? Io temo che poi questi indirizzi verranno applicati in altri campi. Se usassimo gli stessi criteri sulla circolazione stradale, dovremmo adottare delle norme a favore di chi segnala, magari in modo generico, che un certo automobilista ha commesso una irregolarità. Allora per chiunque circoli sulla strada si dovrebbe dimostrare di aver preso delle misure per fare in modo di facilitare la denuncia da parte di chi eventualmente vedesse qualcuno sospetto di commettere un'infrazione stradale. Ma qui veramente abbiamo una roba manicomiale; in confronto il processo di Kafka è una cosa lineare e con le tutte garanzie per l'imputato. Insomma, cerchiamo di tornare alla realtà. realtà. Attenzione, grazie ai cittadini italiani abbiamo il bicameralismo, ma non buttiamolo via, perché se la Camera approva una norma di questo genere e poi noi la lasciamo praticamente immutata, guardate che questa roba diventa legge e causerà gravissimi danni alla pubblica amministrazione. L'unica parte positiva sarà la parte inapplicabile e poi ci porterà verosimilmente, come ha evidenziato il senatore Palma, a una pronuncia della Corte costituzionale. alla pubblica amministrazione e al tessuto produttivo del Paese, che hanno bisogno di poter lavorare per raggiungere i risultati che si prefiggono sia la pubblica amministrazioni che le aziende private, e non di riempire montagne di carta per dimostrare che si è onesti. che si è onesti e che si lavora bene lavorando bene e non commettendo reati. Chi commette reati deve essere punito; chi segnala chi commette dei reati deve essere tutelato, ma non può esserci una alluvione di carte per dimostrare la buona fede o che comunque non c'era malafede. Non Non è possibile una cosa di questo genere. Questo provvedimento è nato - l'ho sottolineato già nella scorsa seduta - per fare una bella conferenza stampa quando si presenterà la legge, dicendo che si è contro la corruzione e ricevendo

emendamento prevede che le disposizioni di questa legge si applichino agli illeciti commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

l'estate scorsa, se è segnalato nel corso dell'anno prossimo (cioè quando la legge sarà in vigore), darà luogo a tutte le tutele previste. Ma io questo

ma qui non si punisce l'evento illecito (notate bene). Vedo che per il senatore Ichino è tutto chiarissimo: se vorrà, prenderà la parola e io sarò felice di ascoltarlo. Qui non si tratta di punire l'atto illecito, in quanto non c'è nessun intervento sull'atto illecito originario, ma si tratta delle tutele verso chi segnala; dunque si suppone che sia quello, però poi c'è il fatto della segretezza. Insomma, qui non si capisce qual è l'applicazione, ma si capisce di sicuro che, nell'ambito dell'indeterminatezza, aumenteranno le misure preventive e difensive da parte di tutti coloro (praticamente tutti) che possono essere colpiti da questa legge. Ricordiamoci che c'è un atto, la multa da 5.000 euro in su, verso coloro che (si deve supporre anche senza saperlo) prendono delle misure di carattere organizzativo che danneggiano qualcuno che abbia segnalato un reato nella pubblica amministrazione, il quale però ha il diritto di restare anonimo e di non essere conosciuto da parte di colui che adotta queste misure organizzative. Dunque, nessuno prenderà più alcuna misura di carattere organizzativo che possa astrattamente danneggiare qualcuno, con una grande efficienza da parte della pubblica amministrazione, che già mi immagino. Credo che tutti sarebbero contenti di migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione oggi, ma in questo modo diventa del tutto sconsigliabile assumere qualunque atto

la norma penale sostanziale, cioè quella che punisce il reato, non certamente le norme volte alla prevenzione e all'intervento di indagine anche su reati o comunque irregolarità commessi commessi in precedenza. Il senatore Malan, che chiaramente faceva riferimento al principio generale *tempus regit actum*, poneva un problema molto serio. un problema molto serio. La normativa prevista in questo disegno di legge, con tutte le tutele che riguardano il lavoratore segnalante, si applica al segnalante che ha segnalato prima dell'entrata in vigore di questa legge e che, per ipotesi, abbia il suo nome già svelato? È una parte della disciplina, che fuoriesce completamente dal principio *tempus regit actum* e che, quindi, pone una situazione di lacuna normativa con riferimento un dato, a mio avviso, molto importante, che è, per l'appunto, la tutela del lavoratore segnalante. Con la conseguenza che il lavoratore che segnalerà del disegno di legge avrà sicuramente le protezioni di cui al presente disegno di legge, protezioni che, a mio avviso, sono molto nebulose invece con riferimento al lavoratore che ha segnalato precedentemente alla sua entrata in vigore.

mentre si capisce quali potrebbero essere i vantaggi che verrebbero a tutta la collettività e all'economia dall'approvazione di questa norma con un corretto funzionamento delle strutture che abbiamo

Risponde - lo sappiamo e lo vedremo con la finanziaria - proponendo di nuovo, sulla scia di quanto aveva fatto il precedente Esecutivo, degli incentivi e degli sgravi fiscali alle imprese perché assumano i ragazzi tra i ignora il dato, che è appunto del 2016 e che dimostra che la politica di incentivi alle imprese non ha funzionato,

I ragazzi sperano di poter investire la loro vita in qualcosa di utile e di importante per il destino dell'intero Paese e non trovano nel lavoro svilito che gli si offre una prospettiva adeguata. Pertanto, vorrei dire ai senatori - ho presentato un'interrogazione sul tema che spero possa avere una qualche attenzione - che la Costituzione prevede una linea alternativa a quella seguita dal Governo Gentiloni Silveri e dal Governo Renzi. Mi riferisco all'articolo 9, che recita: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica». Questa massima della Costituzione è stata seguita nei primi venti anni della Repubblica e non del tutto tradita nei successivi venti. successivamente, è stata completamente abbandonata in nome di un liberismo storico e assolutamente dispersivo di capacità. Oggi c'è un numero enorme di lavoratori precari negli istituti di ricerca costruiti nel primo ventennio della vita repubblicana. Questi precari fuggono all'estero o finiscono con il non essere più degli ottimi ricercatori perché sviliti da una condizione di lavoro inaccettabile. Noi possiamo correggere questa situazione. Propongo che i 300 milioni, anche se pochi, che si possono dedicare a un investimento in finanziaria, siano destinati a stabilizzare i 10.000 precari degli istituti di ricerca del nostro Paese. Diamo la prova che vogliamo investire sul futuro, che vogliamo credere nei nostri giovani e nella loro capacità di rinnovare con il loro lavoro l'intero Paese invece di continuare con gli sgravi e con i regali

una giornalista che indagando tra decine di *file*, carte, numeri e conti correnti era arrivata a delle

La signora Daphne Galizia aveva il fondato sospetto che questo giro di soldi, di tangenti, di corruzione, per cui il suo ultimo *post* appariva quasi disperato, fosse legato al gasdotto TAP,

anche un europarlamentare, Luva Volontè, e ci sono due miliardi di fondi pubblici che arrivano dalla BEI, di cui ricordiamo che il 16 per cento sono soldi italiani. Vogliamo ricordare anche che il Partito Democratico è un forte sostenitore di questo gasdotto, malgrado vi sia una forte opposizione da parte del territorio. Ma Matteo Renzi si è chiuso in un teatro, ha mandato via cittadini inermi e disarmati che volevano semplicemente parlare con lui, ha mandato via universitari, studenti e anche giornalisti onesti, competenti, professionali che volevano solo fargli delle domande, li ha sbattuti fuori e ha continuato a parlare di un tubo che non avrebbe dato fastidio a nessuno, dicendo anche che i comitatini non danno fastidio a nessuno. È saltata in aria una giornalista di cinquantatré anni che lascia il marito e dei figli. Io invito quest'Assemblea e lei, Presidente, a chiedere al Governo di pretendere chiarezza e di non vivere nell'opacità perché il Partito Democratico non ha detto una sola parola su questa storia che è avvenuta, lo ripeto, nel cuore della civile Europa. Presidente, colleghi, vorrei sollecitare l'Esecutivo

aste giudiziarie fallimentari relative al territorio di competenza del tribunale e della procura di Taranto siano in qualche modo pilotate al fine di garantire vantaggi indebiti anche per appartenenti alla magistratura, sempre che l'ipotesi in questione sia verificata. Sappiamo anche che a gennaio 2017 era stata programmata dal Ministero di grazia e giustizia un'ispezione presso il tribunale di Taranto. Questa ispezione dovrebbe essersi conclusa ormai da mesi senza che però sia stata data notizia dell'esito, né siano state date risposte alle due interrogazioni presentate dal Gruppo. da meridionale vicino ai cittadini tarantini, so già che questa città è stata martoriata da una gestione pessima a livello ambientale e sanitario dal gigante ILVA che, di fatto, è un fondo nero per l'economia italiana e soprattutto per la salute di tanti e tanti cittadini. Reputo però che, se a questo dato si deve aggiungere un caso

legali e gli avvocati che si sono esposti denunciando, abbiano necessità di avere risposte. Ricordo che nella vicenda sono coinvolti anche il tribunale e la procura di Potenza che, per competenza, è stata richiamata nelle stesse interrogazioni senza avere tuttavia alcuna risposta. Noi, che siamo considerati i giustizialisti, vogliamo dal Ministero della giustizia delle risposte. Il dubbio,

gestione delle assicurazioni di Roma. Nell'interrogazione, frutto di una serie di documenti pubblici emersi da una fonte sindacale, ponevo una serie di domande

dalla quale emerge con nettezza, e senza possibilità di dubbio, che i temi che avevo posto nell'interrogazione, che facevano apparire opaca la gestione da parte del presidente Sanasi d'Arpe di Assicurazioni di Roma erano del tutto infondati. Ritengo che il sindacato ispettivo sia uno strumento

di Assicurazioni di Roma, professor Sanasi d'Arpe, una correttissima gestione della stessa e credo sia giusto farlo nella sede deputata, che è appunto l'Assemblea.

La seduta è tolta